assistita, già previsto per la seduta di oggi, resta in calendario ma quale ultimo punto, con la clausola «ove concluso dalle Commissioni». Nella seduta di oggi sarà quindi discusso il disegno di legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

ritengo doveroso che in quest'Aula si ricordi una figura di spicco della storia politica e sindacale italiana come quella di Ottaviano Del Turco, scomparso dopo una lunga malattia lo scorso 23 agosto 2024. Ottaviano è stato tra gli esponenti di matrice socialista più in vista della CGIL, dove entra nel turbolento 1968, aderendo alla Federazione dei metalmeccanici (FIOM), per poi diventare nel 1983, all'avvento del Governo Craxi, il numero due della CGIL, prima con Luciano Lama e poi con Antonio Pizzinato e Bruno Trentin. Con Lama Con Lama segretario, vive da protagonista e dall'interno dell'organizzazione tutta la vicenda dell'accordo di san Valentino e la successiva fase referendaria, attestandosi su posizioni riformiste e pertanto opposte alla maggioranza comunista. Vive così da vicino e sulla sua pelle i ritardi e le contraddizioni interne a una certa sinistra, lo scontro tra massimalismo e riformismo che caratterizza la sua storia fin dalle origini. È solo con i tragici e infausti eventi del biennio 1992-1994, con i furori giustizialisti imperanti del tempo, che Del Turco scende nell'agone politico, divenendo l'ultimo segretario nazionale di un PSI ormai inesistente, ridotto al lumicino da una serie di inchieste politiche mirate e ben orchestrate, che non risparmiano il suo *leader* e migliaia di dirigenti e compagni sull'intero territorio nazionale. Sono anni drammatici e di profonda lacerazione nel gruppo dirigente socialista; meno per gli elettori, che nella stragrande maggioranza scelgono in un moto dell'anima di aderire a Forza Italia. Del Turco, invece, prosegue il suo impegno nelle file del ribattezzato centrosinistra, di cui diviene prima deputato nella XII legislatura, poi senatore nella XIII e XIV, ricoprendo anche l'incarico di Ministro delle finanze nel secondo Governo Amato. Tra i fondatori del PD, la scelta di servire la sua terra d'origine, l'Abruzzo, cui era profondamente legato, si rivelò infausta. Eletto governatore nel 2005, sarà investito a metà consiliatura da un'inchiesta giudiziaria dai contorni a dir poco opachi, abbandonato e dimenticato dai suoi stessi compagni di strada in un solo attimo. Una perdita di memoria selettiva che, con dolore, mi spiace aver dovuto constatare anche nei giorni della sua scomparsa. Del Turco è morto sotto il peso della sofferenza e dell'angoscia di una persecuzione giudiziaria che, iniziata nel 2008, l'ha fiaccato nell'anima ancor prima che nel fisico. È stato assolto da accuse infamanti che il tempo ha portato via: assolto dal reato di associazione a delinquere, assolto dal reato di corruzione, assolto dal reato di concussione, assolto dal reato di falso. Reo di una contraddittoria condanna per una presunta induzione indebita, Del Turco ha vissuto

politica avvezza a un'innata subalternità a un certo mondo giudiziario Oggi, nel ricordarlo, non dimentichiamo di denunciare, così come facemmo nei giorni in cui infuriava la bufera, l'ingiustizia di cui è stato vittima, omaggiando la sua memoria, nella speranza che anche questa vicenda possa essere per tutti noi foriera di insegnamenti. Signor Presidente, le chiedo un minuto di silenzio per ricordarlo.

una personalità come Ottaviano Del Turco, che ha speso tutta la sua vita in tutti i ruoli che ha saputo e voluto svolgere al servizio

Placido Rizzotto, una figura mitica del movimento di lotta contro le mafie e per l'emancipazione dei contadini e dei braccianti del Mezzogiorno, che fu ammazzato proprio dalla criminalità. Del Turco ricordò Placido Rizzotto con un'empatia e una totale capacità di vedere in lui un simbolo non solo di tutta la sinistra, ma - io dico - di tutto il Paese democratico antifascista. Infine, non posso dimenticare l'amarezza che tutti noi provammo, e che in primo luogo provò Ottaviano Del Turco, quando, da Presidente della Regione

è stato ed era, in tutti i suoi ruoli, una persona perbene. Non posso dimenticare l'amarezza che provò. Egli pensò che il Partito Democratico, a cui aveva scelto di appartenere, in quei giorni non gli fu vicino. Nei giorni

In tutte queste dichiarazioni c'era la fiducia nella magistratura, lo stupore e l'amarezza per come una persona perbene come Del Turco potesse essere coinvolta, e c'era l'auspicio che questo incubo si chiudesse nel migliore dei Ecco, questo evidentemente provocò una ferita. Del Turco forse avrebbe voluto di più. Eppure in quel momento tenevamo insieme la fiducia nell'onestà nell'onestà personale di Del Turco e nel suo servizio alle istituzioni con il rispetto per l'azione della magistratura, dichiarando poi - ed era scritto nella dichiarazione del segretario - che tutti sono innocenti fino al terzo grado di giudizio. Detto questo, qualsiasi ferita - lo voglio dire qui a nome del nostro Gruppo - non può minimamente cancellare l'importanza, non solo per il sindacato, non solo per la sinistra, ma per il Paese, di una figura limpida come quella di Ottaviano Del Turco.

questa sera siamo in condizione, anche in questo ramo del Parlamento, di poter ricordare la figura di Ottaviano Del Turco. Come Gruppo Italia Viva alla Camera, attraverso il nostro collega Davide Faraone, abbiamo avuto un'iniziativa analoga, ma pensiamo sia giusto e doveroso ricordare in questa occasione una figura così importante, significativa e ricca di elementi che riconducono alla riflessione attuale e alla prospettiva di Ottaviano Del Turco. si sa l'etimologia della parola memoria è quella di conservare traccia: credo che dentro l'esperienza, la storia, le difficoltà e i silenzi che hanno costellato l'esperienza umana di Ottaviano Del Turco ci sia molto di cui conservare traccia, non solo per l'importanza del lavoro che ha saputo e voluto svolgere come sindacalista riformista e come persona che partiva da una terra controversa e difficile come la realtà della montagna abruzzese e che ha saputo diventare, attraverso l'impegno, il lavoro, il sacrificio e lo studio, uno dei punti di riferimento del sindacalismo italiano dapprima, e poi della vita politica, com'è stato ricordato successivamente, come segretario nazionale di un partito, come fondatore di un altro partito e come governatore di una Regione, quella traccia, quella storia e quell'esperienza sono ancora gravide di una serie di domande. Ci sono ancora tanti punti interrogativi che Ottaviano Del Turco lascia dietro di sé e che sarebbe da ignavi non ricordare e non enfatizzare. Come lei ben sa, signor Presidente, c'è una seconda modalità, oltre a quella della memoria, che è quella di ricordare: l'etimologia del ricordo è - letteralmente dal latino - rimettersi nel cuore. cuore. Io vorrei questa sera, rappresentando un Gruppo in questo contesto, esprimere anche un momento personale di ricordo di Ottaviano Del Turco, nel senso etimologico del termine. Quando mi capitò di andare nella sua Collelongo e lui era provato dall'esperienza che la presidente Craxi ha voluto ricordare, mi sono ricordato che c'era un antico, ma giusto e doveroso atteggiamento nella Prima Repubblica: quando si andava nel posto di qualcuno che era stato importante e aveva servito il Paese, prima di andare ad una manifestazione pubblica, si andava ad omaggiarlo in casa, per salutarlo, confrontarsi e raccogliere anche qualche momento di riflessione. Questa sera vorrei rimettere nel cuore quel pomeriggio a Collelongo, davanti a quel camino, con quel sorriso amaro di Ottaviano Del Turco, che credo ci lasci un impegno per portare avanti una battaglia alla quale lui credeva molto, che era il riscatto degli ultimi attraverso il servizio nelle istituzioni repubblicane. Signor Presidente, ringrazio anch'io la senatrice Craxi per aver voluto prendere l'iniziativa e mi associo, a nome di tutto il Gruppo Fratelli d'Italia,

ricordo volentieri la figura di Ottaviano Del Turco, perché è stato uno dei miei primi momenti di attività politica pubblica. Facevo tutt'altro all'epoca e non mi sarei mai sognato di fare politica, ma nell'inchiesta che lo aveva coinvolto qualcosa non mi tornava ed è stato probabilmente uno dei primi processi dove ho preso in mano le carte. In quelle carte traspariva la figura di una persona che non aveva colpe: le accuse che gli venivano rivolte erano chiaramente pretestuose e lacunose. È stato forse uno dei primi momenti in cui, pur essendo egli una persona totalmente lontana dal mio sentire politico, una vicinanza personale mi aveva spinto ad espormi pubblicamente. Ci sono tuttora i miei interventi a sua difesa nei *forum* politici, che all'epoca erano molto frequentati. Penso che la sua storia sia utile, in ogni caso, per essere migliori. Era un periodo di giustizialismo, e un periodo in cui bastava un'accusa per essere immediatamente bollati come criminali o malfattori. Beh, non è così. Ci sono brave persone, ci sono persone che hanno sempre servito la patria con onore e Ottaviano Del Turco era assolutamente una di queste: ha servito le istituzioni ed è stato una persona dignitosa, al di là delle differenze di impostazione politica. Tutti dobbiamo imparare che, quando c'è un'accusa, non necessariamente c'è un colpevole.

dal punto di vista della sua statura politico-sindacale, non posso che riconoscere le cose che qui sono state dette, la figura di una personalità forte, capace

Grazie di cuore. è con profonda commozione che desidero esprimere, a nome mio personale e di tutta l'Assemblea, i sentimenti di affettuosa vicinanza ai familiari e ai colleghi della dottoressa Maria Celentano, che molti di voi hanno conosciuto come consigliere parlamentare in carica, scomparsa ieri dopo una lunga malattia all'età di sessantasei anni, proprio nel giorno nel quale ricorreva il trentottesimo anno di lavoro in Senato. Il suo impegno è stato tenace, tra le altre cose, come portavoce dell'Associazione consiglieri parlamentari, che ha guidato a lungo all'insegna della massima valorizzazione del ruolo del funzionario parlamentare. Ai figli Federica, Emanuele e Rossella va il nostro pensiero commosso, al Segretario Generale e all'Amministrazione tutta del Senato il nostro cordoglio per la perdita di uno dei suoi più validi componenti. In memoria della dottoressa Celentano invito l'Assemblea ad un attimo di cordoglio.

Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata all'esame del disegno di legge di iniziativa governativa di modifica della legge n. 145 del 2016 recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. È un provvedimento di cruciale importanza per il sistema Paese, in quanto risponde alla finalità di rendere il procedimento di autorizzazione al finanziamento delle missioni internazionali italiane più snello e rispondente alla rapida evoluzione del contesto geopolitico internazionale. La relazione illustrativa, allegata al testo, evidenzia come le modifiche introdotte, che peraltro confermano il ruolo centrale del Parlamento nel processo di autorizzazione e di verifica delle missioni stesse, si inseriscono a pieno titolo nel quadro di un più ampio processo di semplificazione introdotto. Tra le novità più rilevanti vi sono: la possibilità di prevedere in anticipo le possibili interoperabilità tra missioni nella stessa area, l'individuazione di forze ad alta e ad altissima prontezza operativa da impiegare all'estero al verificarsi di crisi o situazione di emergenza, prevedendo una procedura accelerata per l'approvazione, la semplificazione della procedura mediante l'eliminazione della previsione dell'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, l'aggiornamento delle tempistiche annuali dal 31 dicembre al 31 gennaio

partecipazione alle diverse missioni internazionali, il Governo possa individuare dei contingenti di forze ad alta o altissima prontezza operativa da impegnare all'estero, previa specifica autorizzazione parlamentare, al verificarsi di situazioni di crisi o di emergenza ovvero al di fuori delle missioni deliberate. La previsione consentirebbe quindi al Governo di poter disporre di un contingente di personale in prontezza operativa da impiegare nel corso dell'anno in caso di crisi o situazione di emergenza non prevedibili al momento dell'adozione della delibera per rafforzare missioni già autorizzate ovvero in Paesi e contesti in cui non vi siano missioni già operative. L'effettivo impiego delle forze è deliberato dal Consiglio dei ministri previa comunicazione al Presidente della Repubblica. La deliberazione prevista viene trasmessa alla Camera che autorizza o nega tale impiego, con appositi atti di indirizzo, entro cinque giorni, con una procedura accelerata rispetto a quella ordinaria. Inoltre, l'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, n. 3, introduce la principale semplificazione procedurale del provvedimento ovvero l'eliminazione della necessità di adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per la ripartizione delle risorse per la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, senza peraltro farne venir meno l'obbligo di una puntuale quantificazione delle risorse finanziarie occorrenti per ciascuna missione. Nel caso di atti di indirizzo parlamentare, volti ad apportare modifiche alla deliberazione sulle missioni internazionali, sarà necessario recepire il contenuto di una nuova deliberazione del Consiglio dei ministri, previa verifica della corrispondente relazione tecnica. Infine - e mi avvio a concludere - l'articolo 2 prevede che le modifiche alla legge n. 145 del 2016 entrino in vigore dal primo giorno dell'anno successivo alla pubblicazione, per evitare che la deliberazione sulle missioni internazionali del medesimo anno sia retta da due discipline diverse.

secondo me, andrebbero auspicabilmente sempre votati all'unanimità. Quando infatti parliamo delle missioni internazionali e del ruolo dell'Italia nel mondo, soprattutto in un settore così delicato come la difesa, credo che non conti l'orientamento del Governo *pro tempore*: un grande Paese si riconosce perché in politica internazionale ha una linea riconoscibile,

con il variare del colore politico del Governo che lo rappresenta in una determinata fase, avendo una collocazione stabile, riconoscibile, riconosciuta, che dà a quel Paese autorevolezza.

essere partecipi della difesa di zone in cui ci sono tensioni o minacce significa in realtà anche essere a presidio della difesa dei nostri valori. Non nascondiamoci dietro un dito: le democrazie liberali in questo momento sono sotto attacco; c'è un disegno molto chiaro che dipinge le nostre democrazie come regimi deboli e volatili in cui è impossibile pianificare a lunga scadenza perché c'è quel "disturbo"

come Stati sui quali non si può fare affidamento o che non hanno la capacità di avere una visione a lunga scadenza. proprio il fatto che la politica sia diventata volubile e che quel posizionamento stabile anche in grandi Paesi - penso per esempio agli Stati Uniti - non sia più così garantito fa sì che molti osservatori internazionali dicano: in quella crisi internazionale non si arriva a una conclusione perché si aspettano le elezioni americane. Quasi a dire che, a seconda di come andranno le elezioni a novembre negli Stati Uniti, le questioni internazionali potrebbero prendere una direzione o un'altra. Penso che questo racconto sia parte di una crisi secondo me non esiziale delle democrazie e credo che abbiamo tutti gli anticorpi per far fronte a questa volubilità, che è un fenomeno relativamente nuovo, ma certo non possiamo non prendere atto e nota del fatto che quelle autocrazie che attaccano i nostri sistemi si fanno evidentemente forza di questa descrizione che naturalmente non ci fa bene. che il ruolo delle nostre Forze armate (e quando dico nostre intendo dire quelle nazionali, ma in genere quelle della NATO) della NATO) oggi non sia soltanto di tipo militare, ma abbia un eminente significato e senso politico. Teniamo conto in particolare di quello che succede nei due scacchieri più caldi, che sono praticamente nel nostro giardino di casa. Penso all'Ucraina, invasa dalla Russia in barba a qualsiasi norma di diritto internazionale, chiaramente in un attacco che non è stato soltanto territoriale, ma è stato un attacco ai nostri valori. Basta sentire le parole non soltanto di Vladimir Putin, ma del patriarca Kirill quando dice che si attacca l'Ucraina per attaccare un modello decadente come quello democratico occidentale. La stessa cosa vale anche, naturalmente, per la crisi per la crisi israelo-palestinese, con tutti i suoi addentellati. Penso, per esempio, al Libano del Sud, alla parte settentrionale di Israele, che è attaccata da tutti i *proxy* iraniani: gli Houthi dallo Yemen e, ovviamente, Hezbollah dal Libano e Hamas dalla striscia di Gaza, anche in un'ottica di sovvertimento dell'unica democrazia che esista in quel quadro. Naturalmente quella è una democrazia e, come tale, imperfetta. Certamente io credo che le scelte del Governo Netanyahu possano e debbano essere criticate, ma senza mai dimenticare qual è il ruolo di quella democrazia e quale siano la funzione, il ruolo, il diritto di Israele di vivere in sicurezza; anzi, il dovere di Israele di esistere e di poterlo fare in sicurezza, anche in quella situazione così complicata. Quando si arriva a discutere di un provvedimento di questo genere, non bisogna nasconderne

infaticabile e anche per il grande prestigio di cui godono ovunque siano state utilizzate. Al di là dei ruoli di maggioranza o opposizione, io credo sia importante fare in modo che le nostre Forze armate, le nostre missioni, siano adeguatamente finanziate e supportate e che le donne e gli uomini che ci rappresentano in questi quadranti così complicati e così difficili possano avere tutti gli strumenti per tenere alti i valori della nostra democrazia e della nostra Repubblica.

Liebenau, che è un'associazione che si occupa di assistenza alle persone portatrici di disabilità. gli studenti della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Innsbruck, che parimenti assistono ai nostri lavori.

Signor Presidente, quella che andremo a breve ad approvare è la ripartizione delle risorse per il fondo per il finanziamento della prosecuzione nel 2024 delle missioni internazionali.

la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante il riparto delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2024. La richiesta ha visto il passaggio in Commissione difesa, per quanto di competenza, e in Commissione bilancio, per la parte finanziaria. Nel 2024, in virtù della situazione di crisi nel quadro intercontinentale, con la crisi mediorientale e in particolare nella Striscia di Gaza e nel Mar Rosso, le Camere hanno effettuato due distinte deliberazioni: una per l'autorizzazione delle nuove missioni, che ha visto l'avvio di tre nuove missioni internazionali per l'anno 2024, e una successiva per la proroga delle missioni in corso che riguarda la proroga, appunto, per l'anno 2024 di quelle già in essere. Oggi, di fatto,

145 del 21 luglio 2016 non si può definire certamente un *iter* snello e non è un *iter* in linea con le richieste attuali, stante la situazione di instabilità mondiale.

una richiesta di modifica, il 25 gennaio, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che va proprio a riformare tale provvedimento è attualmente all'esame del Senato. Il processo di riforma vede un procedimento di autorizzazione e finanziamento delle missioni internazionali italiane sicuramente più snello, con la previsione di una maggiore flessibilità nell'utilizzo degli assetti e delle unità di personale all'interno di missioni appartenenti alla medesima area geografica. Si consente di pre-individuare forze ad alta e altissima prontezza operativa da impiegare all'estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza, e tutto questo in maniera

Di conseguenza, l'*iter* avviato porterà finalmente alla modifica e allo snellimento delle procedure; il Ministro della difesa aveva, già nelle sue linee programmatiche di inizio legislatura, prefissato l'obiettivo di aggiornare il quadro normativo della legge n. necessaria in virtù dell'evoluzione del contesto globale. Pertanto, tale modifica non va solamente ascritta alla minaccia nel Mar Rosso, ma va anche interpretata alla luce di un disgregamento nell'ordine internazionale - abbiamo visto anche l'invasione russa

internazionali, giunto in Senato a febbraio 2024. Si tratta di una proposta legislativa semplice, che guarda alla semplificazione - scusate la ripetizione - di alcuni processi su una tematica estremamente delicata come quella delle missioni internazionali.

decisionale del Parlamento e, quindi, non incide assolutamente sul nostro ruolo di parlamentari. In un momento storico come quello che stiamo vivendo, con due conflitti (quello russo-ucraino e quello israelo-palestinese) la velocità e la semplificazione

Le modifiche si inseriscono in maniera precisa nel quadro più ampio del processo di semplificazione normativa portato avanti dal Governo Meloni. Su un argomento delicato e - lo ripeto - in un tempo dedicato, la semplificazione normativa è ossigeno, è aria fresca; per citare qualcuno,

col Governo Meloni per il grande risultato raggiunto in Europa con la nomina dell'onorevole Fitto a commissario europeo.

vorrei sottolineare il fatto che abbiamo presentato un emendamento abrogativo dell'articolo 1, proprio perché la pensiamo in maniera totalmente diversa da quello che abbiamo finora sentito in Aula, in quanto viviamo in una situazione di grande

nel lavoro emendativo in Commissione il primo degli emendamenti che presentiamo in parte è stato già accettato e penso che ciò sia opportuno. Su uno dei temi centrali, cioè quello della forza di intervento rapido, soprattutto nei teatri in cui si richiede che ci sia un dispiegamento delle nostre forze, di una missione a guida italiana o che integra una missione europea o di un'organizzazione internazionale,

di questo tipo di intervento di emergenza e dell'utilizzo di un canale preferenziale abbreviato. In parte tale emendamento è stato accolto in Commissione; in parte avevamo chiesto di riformulare meglio cosa si intende per urgenza-emergenza, legandolo anche a richieste di organizzazioni internazionali.

relativa alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, non possiamo non sottolineare lo scontro di civiltà in atto. Siamo di fronte a una spaccatura tra quei Paesi che fanno del totalitarismo la loro cifra distintiva e il blocco delle democrazie occidentali che vedono nella libertà il loro valore fondante. Rinunciare a questo impegno per la pace e la libertà dei popoli, abdicare a questo compito gravoso, ma importante, si tradurrebbe in una rinuncia al nostro ruolo, tradendone quei princìpi che contraddistinguono l'Italia. Significherebbe calpestare la nostra tradizione liberale e democratica, arrendersi all'odio di quei sistemi totalitari e oppressivi che purtroppo ancora oggi riescono a sovvertire uno Stato di diritto e a disintegrare la volontà popolare. La nostra credibilità internazionale e la centralità dell'Italia sullo scacchiere internazionale derivano proprio dalla partecipazione alle missioni internazionali; nascono dal sangue e dal sacrificio dei nostri soldati impegnati all'estero. Anche per loro e per quelle generazioni che ci hanno preceduto lottare per la libertà non può essere considerata una scelta di destra o di sinistra. Mi permetterete se, prima di analizzare nel dettaglio questo provvedimento, esprimerò in questa sede un profondo senso di gratitudine alle donne e agli uomini in divisa impegnati nelle missioni militari internazionali: parliamo di migliaia di connazionali che operano con spirito di sacrificio e dedizione in contesti geopolitici complessi, lavorano senza essere esaltati dalla stampa, rischiano la vita a migliaia di chilometri dalle proprie famiglie. Credo che tutti noi, non solo come parlamentari, ma anche come cittadini, dobbiamo essere orgogliosi di quello che fanno. Sono un orgoglio nazionale, una risorsa che mai come oggi va preservata e salvaguardata. In un momento in cui le condizioni di tensione sono spiccate portano un fondamentale contributo, facendosi apprezzare ovunque nel mondo. Noi siamo con questi soldati, i nostri soldati, con i loro valori non discutibili. Com'è noto, la partecipazione italiana alle missioni internazionali viene autorizzata dal Parlamento ai sensi della legge n. 145 del 2016, legge quadro sulle missioni internazionali, che, al di fuori dei casi di dichiarazione dello stato di guerra, si applica per la partecipazione delle Forze armate e delle Forze di polizia, ad ordinamento militare o civile, e dei Corpi civili di pace a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene, comunque istituite in conformità al diritto internazionale. Il disegno di legge in esame, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 25 gennaio, ha la finalità di rendere il procedimento di autorizzazione e finanziamento delle missioni internazionali italiane più snello e rispondente alle rapide evoluzioni del contesto geopolitico internazionale. La norma dunque introduce un elemento di flessibilità nelle deliberazioni con cui il Governo chiede al Parlamento l'autorizzazione per la partecipazione a una missione internazionale, prevedendo in anticipo le possibili interoperabilità tra missioni nella stessa area. In questo modo viene introdotto un elemento di flessibilità nel dispiegamento del personale sui diversi teatri operativi, in virtù dell'evoluzione dei singoli scenari, intervenuti successivamente alle delibere parlamentari. Il personale già operativo sul terreno può essere destinato a rafforzare un'altra missione nella medesima area geografica. Inoltre, il provvedimento prevede che nelle deliberazioni con le quali chiede al Parlamento l'autorizzazione alla partecipazione alle diverse missioni internazionali il Governo possa individuare dei contingenti di forza adatti ad altissima prontezza operativa da impiegare all'estero, previa specifica autorizzazione parlamentare, al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza e, quindi, al di fuori delle missioni deliberate. Questo consentirebbe al Governo di poter disporre di un contingente di personale in prontezza operativa da impiegare nel corso dell'anno, in caso di crisi o situazioni di emergenze non prevedibili al momento dell'adozione della delibera. La norma in esame posticipa la data di presentazione della relazione analitica dal 31 dicembre al 31 gennaio dell'anno successivo. La modifica è motivata dalla circostanza che al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le missioni non sono sempre disponibili tutti gli elementi relativi a loro andamento e ai loro risultati. Infine, il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali è ripartito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, conformemente alla deliberazione del Consiglio dei ministri. La nostra Nazione, fondatrice e non solo membro dell'Unione europea, parte integrante dell'Alleanza atlantica, vuole ribadire, anche attraverso la norma che ci apprestiamo a votare, il suo impegno e la sua adesione a quei valori che ci spingono a partecipare a missioni militari e civili, perché ne va non solo della sicurezza fuori dai nostri confini, ma anche della salvaguardia dell'interesse strategico difensivo sul suolo italiano. Siamo consapevoli che il mantenimento della pace sia un fattore indispensabile per la crescita e lo sviluppo dei singoli Paesi, ma alle volte non bastano le condanne a specifiche aggressioni: bisogna intervenire in maniera diretta per scongiurare effetti destabilizzanti sugli equilibri geopolitici mondiali, crisi come ad esempio quella che colpisce la sicurezza alimentare, che non possiamo sottovalutare. In uno scenario internazionale in costante mutamento, le ricadute dei singoli conflitti amplificano la necessità di un generale riallineamento degli obiettivi strategici, puntando su uno sforzo coordinato per controllare quelle minacce che derivano da più fattori. Il nostro Paese è protagonista all'interno delle coalizioni internazionali, con un'attenzione strategica prioritaria alle regioni del Mediterraneo allargato

più fragili dell'area, in particolare su quelli del Sahel. L'Italia è protagonista delle missioni internazionali con una grande capacità dal punto di vista militare. La nostra Nazione è un attore importante non soltanto nel Mediterraneo allargato, che è il nostro bacino di particolare interesse, ma ormai anche in tutte le aree geopolitiche. L'indirizzo di un Paese come l'Italia, che coniuga la diplomazia all'attività dei nostri militari in tutti i teatri in cui operano, riesce a garantire la tutela della pace e della stabilità. Siamo consapevoli della necessità degli sforzi che, come Paese a guida del G7 (che ha la presidenza di turno del G7), dobbiamo profondere perché si avviino tavoli negoziali. Gli ultimi conflitti hanno scosso profondamente le fondamenta stesse del sistema delle relazioni internazionali costruito nel secondo Dopoguerra. Dobbiamo essere consapevoli che l'Italia mantiene, come caposaldo della propria azione, un multilateralismo imperniato sul sistema delle Nazioni Unite. Non esiste, nei tempi in cui viviamo, una Nazione che possa permettersi di mettere da parte la difesa e le Forze armate. Siamo certamente consapevoli e convinti della necessità di proseguire con le missioni internazionali in corso, nonché con gli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, che sono un elemento fondamentale della politica estera italiana. Solo così si potranno ottenere dei risultati in un contesto che vedrà sicuramente l'Italia vera protagonista. Il popolo italiano non dimenticherà mai ciò che fanno i nostri connazionali all'estero, impegnati in simili contesti per far tacere le armi e risuonare l'arma del dialogo, per un contesto globale che garantisca la sicurezza e la libertà di tutti i popoli.

la sicurezza delle persone e dei nostri cittadini è probabilmente una delle questioni, se non la questione e la funzione più importante cui uno Stato democratico deve assolvere. E quindi discutere delle modalità con le quali si organizza una delle funzioni in grado di garantire la sicurezza dei nostri cittadini, e cioè, nella questione specifica, le modalità con le quali Governo e Parlamento autorizzano le nostre missioni internazionali in un quadro di pace e di accordi bilaterali o di applicazione delle risoluzioni internazionali delle Nazioni Unite, non è certamente un esercizio banale. banale. Questa affermazione di carattere generale deve essere collocata inoltre nella circostanza temporale che noi viviamo

di riordino realizzata otto anni fa, alla quale avevamo convintamente concorso nella definizione di quel percorso legislativo. Questo anche a dimostrare, prima di entrare nel merito, signora Presidente, che - dal nostro punto di vista - le questioni relative alla politica estera, alla politica estera, di difesa e di sicurezza del nostro Paese devono essere il più possibile sottratte a una interpretazione di tipo fazioso o a un utilizzo ai fini di una facile propaganda interna. non solo perché i nostri militari hanno bisogno di sentire dietro di loro, attraverso l'espressione del nostro voto, tutto il popolo italiano *(Applausi)*, ma anche perché, lungo questo versante, la condivisione e lo sforzo di convergenza, che devono esservi tra maggioranza e opposizione, sono la garanzia che sia possibile esplicare al meglio una funzione estremamente delicata che, come tale, non può essere soggetta a questioni di facile polemica interna. Dico di più.

in queste ore il Governo sta costruendo il Piano strutturale di bilancio, che è la modalità con la quale il Governo italiano impegnerà i prossimi sette anni del bilancio del nostro Paese, cioè tutta la legislatura

che non si sta compiendo uno sforzo per venire incontro ad una condivisione di carattere generale, dal momento che si sta costruendo un pilastro che impegna la legislatura attuale e quella successiva. Nella logica della democrazia dell'alternanza, le forze che oggi sono all'opposizione si potrebbero trovare domani a governare, ereditando una misura che non è stata in alcun modo discussa, confrontata e analizzata insieme. Ecco, almeno su questo aspetto, quello delle missioni internazionali, noi siamo dell'opinione che non bisogna compiere un tale errore, proprio per le questioni che ho cercato di ricordare sin qui. Anche perché le evoluzioni che stanno conoscendo le tensioni internazionali impongono sempre più una capacità di risposta adeguata ai tempi. ai tempi. Riflettiamo, per esempio, sul fatto che noi arriviamo ogni anno a licenziare l'autorizzazione parlamentare delle missioni internazionali - quando va bene

velocizzare la capacità di risposta. Pensiamo che sia possibile contemperare le due questioni - l'indirizzo parlamentare, da un lato, e il controllo dell'azione parlamentare, dall'altro con la necessaria assunzione di responsabilità da parte del Governo rispetto ad alcune scelte. Oggi abbiamo un Governo di destra, domani speriamo che questo Governo di destra con le sue forze politiche vada in minoranza, ma il ragionamento è esattamente analogo, perché è il Paese, è la Repubblica che deve essere capace di rispondere adeguatamente in tempi corrispondenti anche alle modalità con le quali altri Paesi a noi alleati, a noi vicini e a noi amici, compiono questo tipo di scelte. Lo dico anche perché, probabilmente, saremo chiamati ulteriormente come sistema Paese a farci carico di ulteriori misure. Se voi puntate sulla mappa geografica già oggi la presenza delle nostre forze sul teatro, potete immaginare plasticamente qual è anche la questione di cui stiamo discutendo. Oggi abbiamo le nostre Forze armate presenti in Bosnia, in Kosovo,

non avevamo condiviso, ma che comunque sono state mantenute perché un Paese serio non fugge di fronte all'esigenza di dover dare delle risposte dal punto di vista della condivisione internazionale. tutta questa descrizione che ho cercato di fare, dimenticando per diversi aspetti anche altre questioni, dimostra quali il ruolo, l'importanza e la strategicità del nostro Paese. Tutti noi auspichiamo, aneliamo e speriamo che ci sia finalmente la capacità di giungere a un cessate il fuoco nelle due grandi realtà complesse che stanno attraversando la tensione internazionale degli ultimi mesi, e cioè l'Ucraina e la Striscia di Gaza. la possibilità di una interposizione di forze nella Striscia di Gaza inevitabilmente richiama l'esigenza di un impegno dei cosiddetti Paesi arabi moderati, il giorno in cui si arriverà - a Dio piacendo e l'uomo volendo - alla possibilità di un cessate il fuoco in terra di Ucraina, è probabile che, attraverso una risoluzione delle organizzazioni internazionali a cui siamo chiamati, ci possa essere anche un impegno del nostro Paese in maniera diretta o indiretta. Come potete è di questo che stiamo parlando e la capacità e l'esigenza di poter avere risposte adeguate in tempi necessari sono direttamente correlate con la nostra capacità di essere presenti nei teatri in maniera omologa e analoga rispetto agli altri *partner* internazionali. Altro è - e concludo, signora Presidente la nostra valutazione rispetto alle modalità con le quali il Governo sta esplicando il proprio ruolo all'interno di quei teatri. Abbiamo notato anche nella visita di ieri che la Presidente del Consiglio - mi riferisco alla visita del Primo ministro britannico - si è sostanzialmente avvitata attorno al noto concetto dell'armatevi e partite. Sappiamo perfettamente che all'interno della maggioranza ci sono delle opinioni divergenti rispetto alle modalità di sostegno dell'Ucraina, ma questa è una questione che affronteremo in un'altra sede. Su questo abbiamo delle opinioni differenti, ma tutto ciò non ci esime dal dire che su operazioni di questa natura le forze temporaneamente temporaneamente di opposizione, che hanno una maturità di Governo e che ritengono attraverso questa esplicazione che potranno tornare al Governo, daranno un voto favorevole.

e in sostanza interviene introducendo modifiche alla legge n. 145 del 2016, una legge quadro che regola la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, con particolare riguardo al procedimento di autorizzazione e finanziamento delle missioni e nello stesso tempo agli scostamenti. Vorrei ora sottolineare un punto. Ho fatto una battuta prima, illustrando l'emendamento soppressivo. In sostanza, si motiva questa scelta come elemento di semplificazione, perché adesso bisogna essere più rapidi nelle decisioni. A noi pare si faccia esattamente il contrario

sono in corso guerre. Perché stabilire che il Parlamento diventa un elemento di freno rispetto a temi così rilevanti, così importanti, così delicati?

Poi si informa al Parlamento, ma quando si informa il Parlamento, dopo novanta giorni, entro tre mesi, potrebbe darsi che il disastro sia già

il Governo ha un'impostazione. Su questo non c'è dubbio. Tutte le maggioranze dovrebbero avere un'impostazione, ma un conto è avere un'impostazione politica, che si riconosce; altro conto è

decise; in altri casi abbiamo dovuto modificarla, ma siamo sempre stati in grado di dare una risposta. Il nostro Paese non si è sottratto a una tale impostazione. Per questo riteniamo davvero che sia un errore pensare di semplificare detta impostazione.

sul teatro sia europeo che mondiale? Oggi noi dovremmo discutere con grande forza, ad esempio, di come interveniamo, in questo caso politicamente, sul genocidio che sta avvenendo a Gaza, in Cisgiordania. Tutti i giorni vediamo decine e decine di civili morti questo è un altro elemento importante. Forse dobbiamo fare una discussione vera su come rilanciare un'operazione di pace

non si può semplificare questa tematica, anzi bisognerebbe aumentare il controllo e la discussione del Parlamento, perché ci dobbiamo assumere le responsabilità di quello che accade. Per questa ragione noi voteremo contro il disegno

colleghi senatori, quella che stiamo vivendo può essere a tutti gli effetti definita un'epoca storica segnata dall'imprevedibilità, nell'ambito della quale, purtroppo, prevalgono sempre più le ragioni delle idiosincrasie rispetto a quelle connaturate al dialogo e alla collaborazione pacifica. Certo, non bisogna mai assuefarsi all'idea che i contorni del mondo si definiscano all'insegna delle crisi, ma occorre anzi adoperarsi ininterrottamente per per cogliere ogni occasione utile al rafforzamento del confronto costruttivo. Il nostro Paese ha contribuito e contribuisce al mantenimento della pace, alla difesa del diritto internazionale, all'opera di prevenzione dei conflitti, al ristabilimento e al rafforzamento delle condizioni della sicurezza, in conformità con i principi della Carta dell'ONU. È una predisposizione alla pace, al dialogo e alla ricerca dei motivi che uniscono più che delle logiche che separano logiche che separano e si articola non soltanto con lo strumento delle operazioni militari di *peacekeeping* e *peacebuilding*, ma anche manovrando la leva della diplomazia culturale, della diplomazia parlamentare e della diplomazia pubblica. È un dato di fatto, però, che nell'attuale contesto globale siano inutilizzabili le categorie interpretative e gli schemi di comprensione del passato. Allora, muovendo da questo presupposto, va detto che il cambio di paradigma nella traiettoria degli equilibri internazionali, dovuto anche al nuovo protagonismo di alcuni *player*, rappresenta un rischio e al tempo stesso l'opportunità per ridefinire alcuni connotati strategici. È in tale scenario che si inserisce questo provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea, che si nutre della primaria finalità di rendere il procedimento di autorizzazione e finanziamento delle missioni internazionali italiane più lineare e rispondente alle rapide evoluzioni dello scenario geopolitico internazionale. Fra le novità più rilevanti che vengono introdotte, va segnalata quella che riconduce alla logica di prevedere in anticipo le possibili interoperabilità fra missioni nella stessa area geografica, in modo da essere in grado di adoperarsi con una maggiore prontezza nell'eventualità di situazioni di crisi o di emergenza, soprattutto nei quadranti di nostro primario interesse (pensiamo proprio al Medio Oriente). Un ulteriore tassello prevede poi la possibilità per il Governo di disporre di contingenti ad alta e ad altissima prontezza operativa da impiegare all'estero, previa specifica autorizzazione parlamentare in caso di crisi o situazione di emergenza per rafforzare impegni già autorizzati. Si tratta di modifiche che si inseriscono a pieno titolo nel quadro di un più ampio processo di semplificazione normativa portato avanti dal Governo, che era necessario, è indispensabile per far fronte allo spirito del tempo e non mina in nessun modo il ruolo centrale del nostro Parlamento. Colleghi senatori, oggi non siamo chiamati a esprimerci su nuovi impegni militari del nostro Paese, ma a prendere atto che occorre confrontarci con uno scenario turbolento in continuo e rapido mutamento. È pertanto necessario che le nostre missioni siano in grado di affrontare e gestire ancora meglio che in passato le evoluzioni che si susseguono incessantemente. L'Italia testimonia ogni giorno di più la sua proiezione internazionale come forza di pace, dialogo e mediazione negoziale; per raggiungere questi obiettivi occorre agire e spendersi sui diversi tavoli, mettendo anche in conto possibili rischi, salvo che non vogliamo condannarci a un isolamento anacronistico e utopico. In ragione di questo profondo convincimento e dell'evoluzione maturata nelle dinamiche internazionali, desidero rinnovare il sentimento di profonda riconoscenza ai nostri militari.

va incontro alle esigenze delle nostre donne e dei nostri uomini in divisa, pertanto annuncio convintamente il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Ritengo ci siano alcune criticità fondamentali che emergono da questa proposta, la prima delle quali riguarda l'ampliamento delle missioni militari internazionali. Con il disegno di legge il Governo si prende la possibilità di inviare forze militari italiane in scenari di crisi anche in assenza di un coinvolgimento diretto dell'Italia o di obblighi internazionali derivanti da trattati. Questa decisione apre la porta a una partecipazione italiana sempre più ampia e indiscriminata in conflitti che potrebbero non riguardarci direttamente. Facciamo l'esempio della crisi ucraina:

il Parlamento deve discutere in cinque giorni (quindi nell'immediatezza, col carico emotivo del momento) se approvare o no la partecipazione a questa missione. Secondo noi il tempo è troppo breve, si rischia appunto, con il carico emotivo del momento, di prendere la decisione sbagliata. Dov'è la necessità di militarizzare ulteriormente la politica estera italiana? Ci si chiede se un Paese come il nostro, che si è sempre distinto per la sua attenzione ai valori umanitari e alla diplomazia, debba davvero assumere un ruolo sempre più interventista. Noi crediamo di no. In secondo luogo, il disegno di legge prevede un minor controllo parlamentare sulle decisioni di invio delle truppe all'estero. Le nuove disposizioni permettono un intervento più flessibile - come ho già citato - da parte dell'Esecutivo, riducendo i tempi del coinvolgimento del Parlamento nelle scelte strategiche militari. Questo, secondo noi, è un *vulnus* per la democrazia. Le scelte che riguardano l'impiego delle nostre Forze armate devono passare sempre attraverso un dibattito compiuto e trasparente in Parlamento, con un confronto chiaro e pubblico sulle reali motivazioni di ogni missione. Ridurre il ruolo del Parlamento in queste decisioni significa ridurre anche il controllo democratico sulle azioni del Governo. Vi è anche un aspetto economico non indifferente. Il costo delle missioni internazionali per il nostro Paese è già molto alto e il presente disegno di legge prevede una gestione molto più flessibile dei fondi, senza però fornire sufficienti garanzie sul loro utilizzo.

dichiarò favorevole rispetto al fatto che le missioni internazionali avessero obiettivi chiari e risultati misurabili, affinché il Parlamento potesse poi decidere in maniera compiuta se prorogare o aumentare i fondi per quelle missioni. Allo stato attuale delle cose, non vedo mai gli obiettivi nelle missioni internazionali e non vedo, a posteriori, un'analisi dei risultati ottenuti, neanche a livello qualitativo. Ci chiediamo se esista un'altra via, diversa e più coerente con i valori che l'Italia dovrebbe promuovere nel mondo. Proponiamo una politica estera basata sul dialogo, sulla cooperazione internazionale e sulla risoluzione pacifica dei conflitti, dei conflitti, che veda l'Italia non solo come protagonista di operazioni militari, ma come un mediatore credibile e rispettato nei tavoli internazionali. diplomazia preventiva dovrebbe essere al centro della nostra azione internazionale: invece di inviare truppe, dovremmo potenziare la nostra rete diplomatica, investire in organismi internazionali come le Nazioni Unite e promuovere accordi di pace. La storia ci insegna che le guerre si evitano con il dialogo, la capacità di sedersi attorno a un tavolo e la negoziazione. Proponiamo inoltre un rafforzamento del nostro impegno in ambito umanitario. Invece di inviare soldati, che pure servono e sono molto stimati, inviamo medici, ingegneri e soccorritori e promuoviamo interventi di ricostruzione post-conflitto e di assistenza alle popolazioni colpite dalla guerra. L'Italia ha una lunga tradizione di cooperazione allo sviluppo: è questa la direzione che dovremmo continuare a seguire. Infine, propongo di investire in una educazione alla pace. Dovremmo promuovere l'educazione ai diritti umani, alla convivenza pacifica e alla risoluzione non violenta dei conflitti. La vera sicurezza internazionale si costruisce anche e anche e soprattutto attraverso la formazione delle nuove generazioni, che devono essere capaci di superare la logica dello scontro e della guerra. un'ultima considerazione. Si dice che in politica la tempistica è tutto e allora provo a evidenziare la vostra tempistica. Oggi in Commissione si sarebbe dovuto votare il parere sul riparto dei fondi delle missioni internazionali, che con questo disegno Ieri è uscito il Documento programmatico pluriennale della Difesa, che incrementa di circa 1,5 miliardi le spese in armamenti e prevede sette miliardi in più per l'acquisto di altri cacciabombardieri F35 nei prossimi anni. arriva questa modifica alla legge sulle missioni, che dà mano libera al Governo per intervenire militarmente ovunque ritenga necessario. Tutto questo dimostra che voi, con buona pace del Parlamento e dei Padri costituenti, che scrissero l'articolo 11 della Costituzione, state militarizzando la nostra politica estera secondo una logica interventista. Per questi motivi, ribadisco il voto contrario del MoVimento 5 Stelle.

soprattutto coloro che, in maniera davvero trasversale, stanno portando avanti temi di grande importanza per il futuro del nostro Paese. Ringrazio anche quelli che fanno un'opposizione prettamente strumentale, perché ci permette di differenziarci e far capire ai cittadini chi veramente, come noi, ha a cuore gli interessi del Paese e chi, invece, utilizza questi strumenti esclusivamente in forma strumentale. Oggi siamo chiamati a discutere dell'importanza della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, un tema di fondamentale importanza non solo per la nostra politica estera,

che combinano operazioni militari, cyberattacchi, disinformazione e utilizzo di forze irregolari. Qualcuno vorrebbe affrontare questi temi sui tavoli dei tecnici e non quelli militari. Queste minacce sono sempre più sofisticate, meno prevedibili e più difficili, evidentemente, da contrastare. Attenzione: le tensioni geopolitiche tradizionali non sono affatto scomparse; anzi, anzi, assistiamo a una recrudescenza dei conflitti regionali e a un aumento dell'aggressività di alcuni attori, anche statali, che cercano di ridefinire gli equilibri di potere, specialmente alle porte del nostro continente e dell'Europa. in Ucraina, ad esempio, è proprio un'evidenza di come i conflitti convenzionali non siano purtroppo relegati al passato, ma rappresentino ancora una minaccia concreta per la stabilità e la sicurezza Tuttavia, le sfide non si limitano solo alle minacce tradizionali. Dicevamo di minacce ibride che combinano elementi militari, economici, tecnologici e informativi e rappresentano una dimensione particolare e anche molto pericolosa della guerra contemporanea, quella che affrontiamo ai giorni nostri. Le operazioni di disinformazione e sabotaggio delle infrastrutture critiche, gli attacchi *cyber* e l'influenza occulta attraverso le forze *proxy* e le milizie irregolari sono diventate parte integrante delle strategie di attori statuali, ma anche non statuali. Tali tattiche sono pensate per destabilizzare le società democratiche e minare la fiducia delle istituzioni internazionali, senza mai sfociare in conflitti diretti che richiedono risposte militari tradizionali. Di fronte a queste sfide, la difesa è tornata assolutamente importante e cruciale. A proposito di Difesa, permettetemi in questa occasione di fare i complimenti al generale Portolano, che è il nuovo Capo di Stato maggiore della Difesa. Complimenti a lui per questo incarico, ma anche un grande in bocca al lupo all'ammiraglio Cavo Dragone per l'importante incarico che andrà a ricoprire all'interno della NATO. non possiamo più permetterci di considerare la sicurezza nazionale e internazionale come un tema secondario, né di lasciare la nostra sicurezza nelle mani di altri, oppure - come dice qualcuno - dei diplomatici. si declina su più fronti: dalla capacità di deterrenza militare alla sicurezza informatica, fino alla protezione delle nostre infrastrutture strategiche e digitali. L'Italia, allora, con la sua partecipazione attiva alle missioni internazionali, dimostra di essere pronta ad affrontare queste minacce su scala - vorrei dire - globale. La nostra presenza in operazioni NATO, ONU e dell'Unione europea è una garanzia di sicurezza per i nostri cittadini, dirlo - per i nostri alleati. Partecipare quindi alle missioni significa non solo proteggere i nostri confini, ma anche intervenire in modo preventivo in quelle aree del mondo dove la stabilità è più fragile, prevenendo l'*escalation* di conflitti che potrebbero coinvolgerci direttamente. Pensiamo, per esempio, al Mediterraneo allargato, una di quelle aree più vicine e critiche per i nostri interessi nazionali: qui la sicurezza marittima è evidentemente minacciata non solo dalla criminalità organizzata e dal traffico di esseri umani, bensì anche dalla competizione geopolitica

In questo contesto, ritengo che l'atlantismo rimanga il pilastro della nostra politica estera e della difesa. La NATO, poi, grazie alla sua capacità di rispondere congiuntamente alle crisi è e deve rimanere l'architrave della sicurezza transatlantica. La nostra partecipazione attiva all'Alleanza atlantica non è solo un dovere, ma è una necessità per garantire la sicurezza dell'Italia e dell'Europa in un contesto globale che, lo abbiamo detto, è sempre più incerto. In questo quadro, è altrettanto essenziale che il nostro sistema di gestione delle missioni internazionali sia all'altezza delle sfide contemporanee. Il provvedimento legislativo che discutiamo rappresenta un passo assolutamente in avanti importante in questa direzione. In conclusione, ritengo di affermare che il mondo sta cambiando; le minacce che dobbiamo affrontare sono sempre più complesse e multidimensionali. In questo contesto l'Italia non può assolutamente permettersi di rimanere in disparte. Partecipare attivamente e in maniera tempestiva

invito tutti (forse inutilmente) a sostenere questo provvedimento legislativo e a confermare con convinzione il ruolo centrale dell'Italia come attore di primo piano nella scena internazionale, difendendo i nostri interessi e quelli della comunità internazionale, in cui crediamo. Per tale ragione, il nostro Gruppo voterà favorevolmente a questo provvedimento.

abbiamo dato una cornice e una legge quadro alle missioni internazionali. Ce n'era bisogno, perché ormai siamo all'estero da tanto tempo, con un numero di missioni che copre praticamente tutti i continenti; le donne e gli uomini della Difesa italiana avevano bisogno di un incardinamento delle proprie missioni, che li coprisse dal punto di vista giuridico ed economico con procedure chiare e che chiamasse il Parlamento e gli organismi competenti a dare linee di indirizzo politico. un atto che desse una cornice a un pezzo della politica estera italiana, che si fa con le iniziative politico-diplomatiche, con le missioni militari, con lo strumento della difesa e con la cooperazione allo sviluppo. Questa legge aveva bisogno oggettivamente di un tagliando, per capire come intervenire su alcuni aspetti procedurali. Abbiamo partecipato al confronto in Commissione affari esteri e difesa, dove alcune nostre proposte sono state accettate e altre no, ma è sicuramente un punto di avanzamento rispetto alle esigenze dei nostri militari, come pure dei Ministeri, nella semplificazione burocratica di alcune procedure e di alcuni passaggi. Ad esempio, già eravamo intervenuti successivamente, nel 2017, per far sì che le delibere che da una parte confermavano e prorogavano missioni già in atto e dall'altra ne individuavano di nuove avessero da subito piena copertura finanziaria, con indicazione degli oneri, dei dispositivi, dei mezzi e del personale e con tabelle che individuavano il costo di ogni singolo intervento, voce per voce. È quindi inevitabile che all'interno di questo provvedimento, di questo tagliando alla legge n. 145, ci siano una semplificazione normativa, ma anche l'eliminazione di un passaggio che portava a nuovi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per il riparto dei fondi fra le missioni, quando invece c'è già tutto, ed è abbastanza chiaro, nelle delibere che prorogano e individuano nuove missioni. Cosa diversa è il controllo che può esercitare il Parlamento, in ogni fase, verificare se siano spese bene o no le risorse per le nostre missioni. C'era un secondo aspetto: una norma che non prendeva atto della situazione sul campo, cioè la possibilità di avere una relazione in tempi ragionevoli alla base delle decisioni che dovevamo prendere e degli atti di indirizzo volti a correggere le finalità operative, politico-diplomatiche e militari delle singole missioni. Si diceva che, per poter

delle Assemblee parlamentari, in modo tale che i nostri militari all'estero abbiano un chiaro indirizzo politico sulle finalità, ma anche sulla valutazione delle singole missioni. Il 31 gennaio è una data congrua.

due dispositivi nazionali nell'ambito di una cooperazione internazionale. Avevamo altresì un'altra operazione di cui abbiamo avuto la guida in alcune fasi, l'operazione europea Eunavfor Atalanta. Eunavfor Atalanta. Ecco, con questa norma garantiamo la possibilità di scambiarsi dispositivi, mezzi navali, aerei e militari, tra un'operazione e l'altra, rendendo più flessibile

L'altra innovazione è più delicata, perché ha bisogno di pesi, contrappesi e anche di controlli adeguati dal punto di vista parlamentare: è quella di un canale preferenziale in caso di emergenza e urgenza e di gravi crisi internazionali. Si prevede una procedura di cinque giorni per poter deliberare una nuova missione internazionale.

una missione con i caratteri dell'urgenza e dell'emergenza per una grave crisi internazionale. Abbiamo apprezzato questo passaggio. Noi avremmo anche inserito un passaggio con il Consiglio supremo di difesa, mentre qui si parla solo della previa comunicazione al Capo dello Stato che, lo ricordo, è anche comandante delle Forze armate. Da questo Da questo punto di vista, noi avremmo previsto un passaggio nel Consiglio supremo di difesa. È vero che il Presidente della Repubblica può essere coinvolto in qualsiasi momento, ma prevederlo sarebbe stato una procedura più lineare, coerente e in qualche modo rispettosa del ruolo del Capo dello Stato. Comprendiamo però che in una fase di grande cambiamento nelle relazioni internazionali e nella capacità di essere operativi e di intervenire prontamente in maniera immediata in questi teatri di crisi possa avere senso, in linea con quanto si sta facendo anche a livello europeo, con la *strategic compass*, con la nuova bussola strategica, che ha portato a individuare proprio una forza

della nostra proiezione all'estero dal punto di vista militare, con le missioni internazionali di *peacekeeping*, al fine di avere uno strumento in più che avrà bisogno chiaramente sempre degli opportuni contrappesi, cioè dei controlli parlamentari e degli atti di indirizzo politico. Quindi, nonostante alcune perplessità e criticità che abbiamo messo in evidenza, su cui continueremo a lavorare, pensiamo che queste modifiche rappresentino un passo in avanti che dà certezza alle nostre Forze armate, che approfittiamo per ringraziare da parte del Partito Democratico per il ruolo e il lavoro che svolgono in giro per il mondo in teatri sempre più complessi.

per far sì che la loro capacità di rappresentarci al meglio all'estero potesse essere oggettivamente fondata su una unanimità espressa anche da un voto parlamentare.

quando sembra che il Governo non sia tale: andiamoci a leggere l'attuale Costituzione e speriamo che i prossimi Governi, con una forma anche differente a seguito di una modifica costituzionale, abbiano un ancor maggiore fondamento democratico. Stavo dicendo che il Parlamento

Governo. Parlare di aumento di spese militari quando l'accordo sul 2 per cento con la NATO l'ha preso colui che oggi è *leader* del MoVimento 5 Stelle e che all'epoca era Presidente del Consiglio dei ministri mi sembra un pochino ipocrita, quando l'attuale Ministro della difesa,

dei nostri militari in Ucraina: in quel caso, saremmo fuori da una missione internazionale; saremmo nel caso previsto dall'articolo 78 della Costituzione, che Dio non voglia mai dovessimo applicare. Quindi non c'entra assolutamente nulla; è un esempio completamente sbagliato e infondato. Oggi, in uno scenario internazionale complesso, sono stati giustamente citati più volte i conflitti di cui anche mediaticamente più si parla, come quello a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina o il tema del Medio Oriente e dell'eterno conflitto tra Israele e il popolo palestinese. Ci sono inoltre dei focolai, forse più vicini a noi da un punto di vista geografico, non solo è giusto attenzionare, ma su cui dobbiamo accendere una luce per evitare che possano generarsi effetti a catena che potrebbero dare dare risultati devastanti: penso alla vicenda del Nagorno-Karabakh tra Armenia e Azerbaijan; penso a tutto ciò che ancora cuoce sotto le ceneri tra il Kosovo e la Serbia nell'ambito della questione balcanica; penso a una serie di situazioni che pongono quel pezzo orientale di Occidente - non è un ossimoro, ma un paradosso geografico - che noi rappresentiamo

che cosa votarono nel 2016 alla Camera dei deputati nove rappresentanti di Fratelli d'Italia, ma credo che aver avuto il coraggio di imporre o proporre una legge quadro sulle missioni internazionali fosse qualcosa di sicuramente giusto. Come però lei stesso ha riconosciuto, è chiaro che questa legge aveva bisogno di un tagliando, perché, in questi otto anni, evidentemente

i nostri militari in giro per il mondo in missioni internazionali non fanno azioni di guerra. I nostri militari nel mondo in missioni internazionali costruiscono ponti e strade con il Genio; intervengono da un punto di vista medico, assistenziale e sanitario; compiono opere di vera socialità nei confronti delle popolazioni colpite da contesti interni o internazionali complicati. Quindi, anche su questo, cerchiamo di raccontare realmente quello che fa

aumentano la saldatura tra lo Stato che ospita temporaneamente i militari italiani e l'Italia, che hanno sviluppi diplomatici, a volte anche economici, grazie appunto alla credibilità che i nostri militari italiani ci conferiscono all'estero.

rivoluzionaria, ma credo sia un passettino avanti verso la sburocratizzazione di una Nazione in cui, anche in questo campo, c'era bisogno di intervenire. Ci potrà dare in più, in alcune occasioni particolari, per essere tempestivi, quindi è evidente che il Gruppo Fratelli d'Italia voterà convintamente a favore rispetto a questa normativa.

il 14 settembre, sulla base del nostro calendario, cadeva il secondo anniversario dell'omicidio di Mahsa Amini. Ricorderete la ragazza iraniana di origine curda, che fu picchiata e poi arrestata dalla polizia morale perché non indossava il velo in conformità alla legge e qualche ricciolo di capelli era visibile. Da quella morte è nato un movimento, «Donna, vita, libertà» a cui credo noi tutti dovremmo guardare con attenzione ed anche inchinarci per la forza straordinaria delle giovani e dei giovani iraniani che hanno continuato a riempire le piazze, a manifestare comportamenti di libertà, a chiedere libertà e democrazia nel loro Paese. Nei giorni scorsi, in particolare nella notte di domenica, la repressione del regime iraniano è stata fortissima, in particolare nelle zone del Kurdistan dove hanno avuto luogo proteste che ricordavano, anche con lo sciopero generale, la morte di Mahsa Amini. L'Europa e l'Italia non hanno fatto tutto quello che si poteva fare per sostenere «Donna, vita, libertà», non l'hanno fatto non dichiarando corpo terroristico il corpo delle Guardie della rivoluzione, quella famosa polizia morale che ammazza;

portare solidarietà a persone che rischiavano la condanna a morte in Iran, ritorno sull'argomento parlando del messaggio che ha mandato dal carcere di Evin la premio Nobel Narges Mohammadi, da lungo tempo, nonostante le sue condizioni di salute, nonostante lo sciopero della fame, nonostante la prigionia che continua, manda dei messaggi. Quello che ci ha mandato, insieme a tutta la rete delle associazioni, è un messaggio che credo sia importante con il quale chiede chiede che si criminalizzi l'*apartheid* di genere. Non è un'affermazione come un'altra, ma significa chiedere all'ONU innanzitutto, ma a tutti i Paesi, di far sì che l'*apartheid* di genere diventi un crimine internazionale e come tale combattibile e contrastabile, che parte da un punto fondamentale: quando si dice che le donne devono sottostare a certi comportamenti, che, come in Afghanistan, non possono andare a scuola, non possono uscire, non possono cantare, non possono lavorare, quando si determina una condizione che, appunto, dobbiamo definire di *apartheid*, non c'è democrazia. Il tema non è solo pensare alla democrazia per quei Paesi, ma è avere il coraggio di riconoscere che, se ci sono zone dove l'*apartheid* di genere è in funzione, questo determina un arretramento per tutte le donne del mondo. Credo un Paese come il nostro debba invece innanzitutto sentire come sorelle sia le donne iraniane, sia le donne afgane. ringrazio, senatrice Camusso, per aver posto all'attenzione di questa Assemblea il tema dell'universalità dei diritti umani e della stretta connessione con qualsiasi azione e attività di politica estera.

piange la scomparsa di Caterina Valente, cantante, attrice, icona internazionale, che ha lasciato un segno indelebile nella storia del panorama musicale mondiale. Era di origine italo francese, nata a Parigi da famiglia italiana, si è spenta il 9 settembre, all'età di 93 anni, a Lugano, in Svizzera. Ha vissuto una carriera artistica lunga, poliedrica e di grande successo. Era nata a Parigi nel 1931 ed era figlia d'arte, proveniva da una famiglia italiana di artisti d'avanspettacolo. Il padre Giuseppe era originario di San Biagio Saracinisco, in provincia di Frosinone, all'ombra delle Mainarde nel Lazio, ed era un noto fisarmonicista. La madre, invece, Maria Siri, era un'attrice e una musicista polistrumentista, nonché ballerina, nata a Roma da famiglia genovese. Caterina iniziò a esibirsi in teatro già da bambina, insieme ai tre fratelli, e si costruì poi una carriera straordinaria che l'ha portata al successo internazionale a partire dagli anni Cinquanta, come cantante, attrice, chitarrista e ballerina. Seppe conquistare il pubblico mondiale non solo con la sua voce inconfondibile, ma anche con la sua versatilità artistica, spaziando dalla musica al cinema e alla televisione. Caterina ha costituito nel Novecento l'esempio paradigmatico di un'artista cosmopolita, anche a seguito delle sue scelte di vita. come detto, nata a Parigi, ma si sposò in prime nozze con un tedesco e in seconde con un britannico, vinse premi internazionali, ebbe un pubblico affezionato in ogni continente; incise oltre 1.500 brani musicali in tredici lingue diverse, di cui almeno Il suo debutto su piccolo schermo italiano è avvenuto nel 1959 grazie a Mario Riva e alla trasmissione «Il Musichiere».

La grandissima Mina in un'intervista disse di lei: Caterina Valente, che io chiamo maestra, è una musicista pazzesca e, come voce e come padronanza, rimane la più forte. Credo quindi che sia una buona cosa ricordarla in quest'Aula come una grande artista che ha onorato l'Italia. *(Applausi)*.